Quanto alla considerazione di metodo, qui siamo tutti ben consapevoli da più di una settimana che la discussione si concluderà con un voto di fiducia,

sulla eccezionale facoltà legislativa che la Costituzione assegna al Governo, vale a dire la discussione e la votazione degli emendamenti. Sarebbe stato molto meno ipocrita e molto più serio da parte del Governo annunciare sin dall'inizio della settimana questa sua determinazione,

Conla finanziaria del 2006 il Presidente del Consiglio ha dimostrato quanto quella sua dichiarazione fosse una falsità, un inganno per gli italiani, ma il metodo del provvedimento è quello tipico della sinistra per la quale si stanga un Paese con le tasse per poi redistribuire a qualcuno una mancia, pensando in questo modo di recuperare in qualche misura il consenso elettorale. Non soltanto perché si dovrà poi procedere ad un voto di fiducia, ma per respingere questo metodo che l'Italia intera rifiuta e

fondare la propria politica economica sulle menzogne e sperare di recuperare credibilità con qualche mancia. *(Applausi Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo «L'isola del tesoro» di Stevenson, ecco «L'isola del tesoretto» di Prodi. Non si tratta, come sapete, di un racconto avventuroso, bensì di un decreto governativo recante disposizioni cosiddette urgenti in materia finanziaria, che il Senato è oggi chiamato a discutere e a convertire in legge. È quindi un documento burocratico che non può certo possedere la vitale grandezza del famoso romanzo, a cominciare dalla statura degli stessi protagonisti: vogliamo forse mettere la feroce simpatia canagliesca di un Long John Silver con la rassegnata prudenza professorale di Padoa-Schioppa? Non si può! Resta però la singolare analogia tra i due testi, considerato che in entrambi si parla di un misterioso tesoro, della sua faticosa ricerca e dell'accanita lotta per accaparrarselo e dividerselo. Che poi tutto questo non abbia molto a che vedere con una seria politica economica è purtroppo un altro discorso, ma chiedere serietà al Governo Prodi, che pur era nato con la presunzione di portarla al potere, sarebbe come chiedere ai pirati dei Caraibi - tanto per rimanere in argomento - di rinunciare al rhum. È semplicemente impossibile. L'assenza totale di serietà caratterizza peraltro questo decreto-legge, così come la vicenda che lo ha originato. Tutto ha inizio lo scorso anno, al momento del varo del DPEF, quando il Ministro dell'economia e delle finanze affermò che la situazione economica e finanziaria peggiore di quella del 1992 e che il debito pubblico era talmente fuori controllo da costringere il Governo alla predisposizione di una pesantissima legge finanziaria, tutta tasse. Una tesi che verrà poi smentita dagli accadimenti successivi che, anzi, riveleranno come il presunto dissesto finanziario causato dal Governo Berlusconi si sia, al contrario, tramutato in un virtuoso extragettito da maggiori entrate fiscali. Ciò è tanto vero che su questo eccezionale extragettito nasce immediatamente, all'interno del centro-sinistra, l'interessata leggenda del tesoretto, che già nella terminologia indica più un bottino da spartire e distribuire secondo criteri di banda che non una massa di risorse da impiegare razionalmente secondo una logica di politica economica. Non a caso, il Governo deciderà di rimanere sordo agli appelli di Bankitalia, di Bruxelles e del Fondo Monetario Internazionale, per destinare - col presente atto - una consistente parte di tali risorse alla spesa corrente, anziché al risanamento dei conti pubblici, col risultato di incrementare la perversa spirale fatta di più tasse, più spesa corrente, più debito. L'impressione è che la leggenda del tesoretto sia servita soprattutto a coprire il ritorno all'antica politica della spesa: intesa quale elargizione di contributi (sia pur minimi) in tutte le direzioni, senza alcun criterio ordinatore. È come se, in pratica, il Governo avesse definitivamente abbandonato ogni idea di programmazione, affidandone il ricordo all'ultima versione crepuscolare contenuta nel DPEF approvato la settimana scorsa. Del resto, il testo del decreto-legge in corso di conversione appare in netta contraddizione con le indicazioni e i princìpi dello stesso DPEF. Esso si pone contro l'obiettivo dell'equità, perché disperde circa 7 miliardi di euro in una spesa a pioggia senza strategia alcuna, se non quella di un maldestro quanto modesto tentativo di limitare i danni arrecati dal Governo con la finanziaria e il decreto Visco-Bersani, la qual cosa è, ad esempio, particolarmente evidente negli interventi riparatori e nelle misure tampone previste per la scuola, l'università e la cultura. Ma è anche contro l'obiettivo del risanamento, perché l'aumento di spesa, da esso causato, viene finanziato attraverso un aumento del *deficit*, tanto da indurre il Governo a correggere il *deficit* «concordato» con l'Unione Europea, portandolo dal 2,1 al 2,5 per cento del PIL. Ed è infine contro l'obiettivo della crescita, perché invece di cogliere l'occasione di un positivo andamento dell'economia per sostenerla e consolidarla accelerando il risanamento dei conti pubblici, finisce col lasciare inalterato il gravame del debito pubblico, ipotecando così ulteriori possibilità di sviluppo. Si può, certo, governare in *deficit*, ma a patto di spendere per le riforme strutturali, non per la spesa corrente. La verità è che la politica del Governo si riduce alla mera gestione del presente o meglio alla programmazione dell'immobilismo, il cui costo economico e sociale viene cinicamente scaricato sull'Italia del futuro.

stiamo o meglio il Governo sta perdendo una straordinaria occasione che aveva per dare un grandissimo impulso all'economia del Paese. Aveva annunciato con la finanziaria 2007 una stagione di rigore; tutti ci siamo chiesti se era il caso di inasprire così la pressione fiscale, dal momento che le necessità erano inferiori a quello che la manovra dell'anno scorso aveva previsto, ma ci fu detto che era troppo importante il risanamento dei conti pubblici. Il Paese era chiamato a grandissimi sacrifici in ragione del fatto si sarebbe leggermente appianata quella grande montagna di debito che sta sotto un lenzuolo e apparentemente non si vede, ma che fa la differenza tra l'Italia e il resto dei Paesi europei. Con che criterio affrontiamo una stagione in cui, in controtendenza, non c'è bisogno di chiedere sacrifici, ma c'è la possibilità di realizzare un intervento straordinario, perché si ha da una parte un qualcosa che non si era preventivato di avere? Tutti si aspettavano la medesima logica con cui questo Governo ha approcciato con il Paese: estremo rigore, accantonamento il più possibile, anche perché

con meno debito c'è meno necessità di farvi fronte per il Paese, per il sistema istituzionale e governativo; si sarebbe potuta abbassare la pressione fiscale e, abbassando la pressione fiscale, rimaneva in tasca qualcosa in più alle famiglie oltre che alle imprese. Rimanendo qualcosa in più in tasca alle famiglie, si sarebbero rilanciati necessariamente i consumi, dando maggiore vigore all'economia; le stesse imprese con una pressione fiscale più adeguata avrebbero messo in ciclo

risulta che i quattro distretti del tessile italiano hanno più addetti, complessivamente, di BMW e del gruppo Royal Shell; i 10 distretti italiani del mobile occupano più persone di Coca Cola e dell'Oréal, grandi colossi internazionali, i sette distretti italiani dei metalli hanno più occupati della Bayer, i sette distretti italiani delle pelli e delle calzature

Questi sono i gruppi italiani. La nostra piccola e media impresa riesce a reggere e, in un momento di crisi, è la risposta economica del Paese. Di fronte a questa necessità, a questa alzata di scudi, a questa chiamata in corresponsabilità di tutto il sistema istituzionale, il Governo fa capire al sistema delle imprese che non gliene importa assolutamente nulla,

una cifra non considerevole, quasi 5 miliardi di euro, senza una *ratio*, senza un principio ispiratore che faccia capire che tipo di manovra fiscale è questa, di che tipo di manovra economica

Se si potesse usare il termine azione criminale,

Signor Presidente, l'Atto Senato n. 1739 al nostro esame, al di là di tutte le considerazioni legittimamente poste alcune delle quali degne di attenzione e di considerazione positiva, trae origine dall'operazione tentata con la finanziaria 2007, il cui risultato era certamente auspicabile, ma non affatto scontato. è stato possibile grazie ad un'azione di Governo che ha coniugato il rigore verso la politica di contenimento e di controllo della spesa pubblica e il recupero di parte dell'evasione fiscale con l'attenzione, anche se ancora parziale, verso le fasce più deboli e le nuove emergenze sociali. Infatti, gli andamenti di finanza pubblica hanno evidenziato un miglioramento dei conti pubblici in termini sia di saldo netto della finanziaria che di indebitamento netto, che nel 2006 è diminuito di 1,7 punti percentuali grazie ad un aumento delle entrate tributarie di circa 1,6 punti percentuali di PIL, mentre la spesa primaria corrente è rimasta pressoché invariata. Ritengo utile ricordare che l'indebitamento netto certificato, ereditato da questo Governo, ammontava al 4,1 per cento e che la spesa primaria corrente alla fine dei cinque anni dei precedenti Governi di centro-destra

Invece, il maggiore gettito è dipeso dal fatto che le imprese, in assenza di una politica di condoni, hanno riportato il proprio fatturato al Il miglioramento dei conti pubblici è da ascrivere, sostanzialmente, al migliore andamento del gettito tributario. Infatti, la nostra strategia di contrasto all'evasione fiscale ha condotto ad un mutamento delle aspettative e a un diverso atteggiamento dei contribuenti nei confronti del fisco. Come ricordato dal vice ministro Visco nel corso dell'audizione di ieri in Commissione bilancio, l'annuncio che non vi saranno più condoni ha reso chiaro che gli evasori La riorganizzazione della macchina dei controlli ha segnalato che la probabilità di essere accertati è reale e significativa; una serie di interventi legislativi ha in parte chiuso alcuni dei canali più evidenti di evasione fiscale, penso per esempio al settore immobiliare o all'importazione intracomunitaria; le modifiche intervenute e che interverranno negli studi di settore migliorano il rapporto tra amministrazione fiscale e imprese. I risultati finora raggiunti sono significativi. Nel 2006 le entrate della Pubblica amministrazione sono cresciute del 9,6 per cento, al di sopra della crescita nominale del prodotto interno lordo, che è stata del 3,7 le entrate del bilancio dello Stato sono aumentate di 35,8 miliardi di euro rispetto al 2005 e più del 30 per cento di questo aumento non è ciclico, ma strutturale ed è legato, appunto, ad un'efficace ed efficiente lotta all'evasione. La crescita del gettito dell'IVA, infatti, ne è l'esempio più evidente: è aumentato del 10 per cento il numero degli accertamenti sui contribuenti con crediti di IVA e l'IVA evasa accertata è cresciuta del 33 Anche l'efficienza della riscossione sta aumentando: nel primo trimestre del 2007 la riscossione dei ruoli, cioè le imposte accertate e dovute, è aumentata del 90 per cento rispetto al 2006; la riscossione diversa dai ruoli è aumentata del 23 per cento; le verifiche ed i controlli mirati nei confronti delle grandi imprese sono aumentati rispetto al 2006 del 21 per cento, con una crescita constatata del 200 Gli accertamenti nei confronti delle società di capitali sono aumentati del 7,4 per cento, con una maggior imposta accertata del 41 per non parlare dei risultati positivi per effetto del decentramento del catasto e delle attività delle Agenzie del demanio. Tutto questo lo si sta facendo per contrastare un'evasione fiscale che in Italia è quasi doppia rispetto a quella della Francia, della Germania, del Regno Unito e quattro volte superiore a quella dell'Austria, dell'Irlanda e dell'Olanda.

In Italia si nascondono al fisco circa 17-18 punti percentuali del PIL, pari a circa 230-245 miliardi di euro (fonte

Con l'evasione si perdono circa sette punti percentuali di PIL in mancate entrate, ogni anno 100 miliardi di euro. Ecco perché è importante l'azione volta a recuperare elusione ed evasione fiscale. Controllare l'evasione e l'elusione è una necessità economica imprescindibile, oltre che un dovere civico e un obbligo morale. Lo sforzo di politica fiscale del Governo continua a dare esiti positivi sulle entrate dei primi mesi del 2007, il che conferma il carattere parzialmente strutturale degli interventi. Infatti, con il primo semestre 2007 si stima una crescita delle entrate di circa il 6 per cento, chiaramente al di sopra della crescita economica che finora si attesta al 4 per cento nominale del PIL. Questi risultati fanno supporre per il 2007 un maggior gettito rispetto alla stessa previsione del DPEF 2008-2011 di almeno 2 miliardi, quindi, oltre 5 miliardi di euro in più rispetto a quanto indicato nella relazione unificata di marzo e di circa 11 miliardi di euro in più rispetto all'obiettivo sottostante alla legge finanziaria scorsa. Tali risultati sono possibili, appunto, grazie alla maggior crescita del PIL nominale e ad un recupero dell'evasione superiore a quanto previsto. Ciò rende possibile l'obiettivo previsto ed indicato nella legge finanziaria 2007 di ridurre il carico fiscale su famiglie ed imprese. Presidente, ho voluto ricordare tutto ciò non perché io e il mio Gruppo abbiamo una particolare attenzione alle politiche impositive o repressive; come è noto noi abbiamo invece una propensione culturale che ci porta a guardare con attenzione alle politiche redistributive in grado di realizzare giustizia sociale, estendere e rafforzare la rete dei diritti, combattere il lavoro nero, stabilizzare e superare quello precario, tutelare l'ambiente e le politiche di solidarietà interna ed internazionale. ciò per rendere chiaro che le maggiori entrate per l'anno 2007 iscritte in bilancio con l'assestamento del 2007, di cui ci occupiamo, appunto, con l'Atto Senato al nostro esame sono il risultato di politiche tenacemente perseguite, i cui risultati positivi si cominciano ora a riscontrare. Occupandoci dell'articolato del provvedimento, occorre innanzitutto far rilevare che con questo decreto il Governo intende assolti gli impegni, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria 2007, che prevedeva che le maggiori entrate tributarie, che si realizzavano nel corso dell'anno, rispetto alle previsioni, siano prioritariamente destinate

che parzialmente lo sono - vanno destinate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di equità fiscale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basso. Queste è quello che si comincia a fare con il decreto al nostro esame. Con l'articolo 5, nei commi da 1 a 4, infatti, si dispongono gli aumenti per le pensioni minime ai soggetti con età pari o superiore ai 64 anni. Si stima che gli interessati nel 2008 siano 3.050.000 cittadini, prevedendo la corresponsione delle somme previste già a partire dal 2007. Con il comma 5, dell'articolo 5, invece, si dispone l'aumento delle maggiorazioni delle maggiorazioni sociali legate in particolare ad invalidi civili, ciechi e sordomuti. 290.000 sono i soggetti interessati. Con il comma 6, sempre dell'articolo 5, si prevede la rivalutazione dei trattamenti pensionistici sulla base di un meccanismo legato ai prezzi, per le pensioni previdenziali, attraverso l'applicazione di indici di rivalutazione. Il comma 8, sempre dell'articolo 5, costituisce un fondo per agevolare il riscatto ai fini pensionistici del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici. Inoltre, nel decreto al nostro esame, di particolare rilievo, sono le norme previste in materia di studi di settore, in coerenza con quanto indicato nella mozione presentata dal centro-sinistra ed approvata dal Senato, che prevedono, in accordo con le categorie interessate, che gli indici di normalità economica avranno natura sperimentale e valore di presunzione semplice fino all'elaborazione e revisione degli studi di settore e e che non potrà scattare più l'accertamento automatico se il risultato cui è pervenuta l'amministrazione derivano dall'applicazione di nuovi indici. Rimane aperta la questione - lo sappiamo - della retroattività Ma nel frattempo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che anticipa la possibilità di adeguarsi anche al minimo previsto dagli studi di settore, purché congrui con il riferimento ai ricavi. Il decreto contiene anche norme importanti per gli enti locali ed, in particolare, per quelli virtuosi, quali la maggiorazione della quota di avanzo di gestione che gli enti locali potranno utilizzare e le nuove norme in materia di rispetto del Patto di stabilità interno; e ancora il Fondo per l'acquisizione di beni e servizi per investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. La semplificazione per la concessione di incentivi alle imprese in materia di crisi di imprese (articolo 8-*bis*) sblocca le somme della legge n. 488 per circa 2,3 miliardi di euro; le norme in materia di cooperazione e di sviluppo (10 miliardi di euro), i trasferimenti alle imprese pubbliche (articolo 8): 250 milioni di euro per il 2007 a favore delle Ferrovie dello Stato, delle Poste italiane, dell'ENAS e dell'ENAV; la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università (180 milioni di euro per il 2007), lo sblocco di riserve vincolate alle quote del TFR delle imprese con più di 500 dipendenti, le norme a sostegno dell'economia ittica, cui viene esteso il credito di imposta. Si tratta di 200.000 euro nel 2008. Come si vede, signor Presidente, si tratta di provvedimenti positivi che vanno nella direzione giusta, in coerenza con le indicazioni della legge finanziaria e con la risoluzione di maggioranza relativa al DPEF 2008-2011, che abbiamo la settimana scorsa approvato. Per queste ragioni, auspicando quindi che anche le altre norme contenute nell'Atto Senato n. 1485 e non contenute nel presente provvedimento vengano recuperate, esprimo il consenso e l'apprezzamento del Gruppo Sinistra democratica al presente provvedimento, annunciando il voto favorevole allo stesso.

da un'economia totalmente falsata. L'Italia ha resistito ed è stata accreditata in Europa,

di questa importanza. Ma Padoa-Schioppa ha altro da fare; credo fosse pochi giorni fa a Viareggio o a Cortina d'Ampezzo, con un bel pulloverino sulle spalle a discutere e ad insultare il presidente Berlusconi,

vanno da Nord a Sud in ugual misura. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ha ben detto il collega Strano: c'è un'unità nel Paese come forse non c'è mai stata. C'è unità a considerare questo provvedimento come un provvedimento farsa, un provvedimento burletta. Non lo diciamo noi, poveri rappresentanti del popolo e sicuramente non nominati dall'alto, ma lo dice un tal Draghi: «È sparito il tesoretto, l'extragettito non c'e più» e poi un certo Gioacchino Almunia, sicuramente un pericolosissimo conservatore, che afferma: «Gli sforzi correttivi dell'Italia per ridurre il disavanzo e il taglio del *deficit* prefigurato nel 2008 non sono all'altezza degli obiettivi». Ma lo dicono anche pericolosissimi reazionari come Francesco Giavazzi, Luigi Spaventa ed altri economisti, che dicono una sola cosa: questo provvedimento non è coperto. Allora, noi pensiamo che non si possa scherzare con le speranze Non si può raccontare per un anno che anche con il freddo e con la nebbia c'era qualcuno che dava dei numeri.

Quindi, fa un progetto per il futuro, investe per il futuro. Ma qui, lo ripeto, stiamo giocando con le speranze degli italiani e dei padani a cui avete promesso che aumenterete le pensioni. Ebbene, sì,

e l'aumento, sempre per questa piccola platea, sarà di 12 euro al mese: meno di un caffè ogni due giorni. Per carità, è sempre meglio di niente; però quando si va a parlare, così come avete fatto, di redistribuzione, di equità, di stato sociale e quant'altro, dovremmo anche considerare che questo provvedimento alla fine non solo non soddisfa nessuno, ma anzi sta scontentando tutti. E adesso, aspettiamo che il

schierati contro, su cui avevate lanciato dei proclami. Quando noi pensavamo di consentire l'accesso al credito ai giovani, giovani, istituendo un fondo per dare le garanzie ai giovani perché potessero comprarsi la casa, voi avete detto di no, e venne stralciato dalla Corte costituzionale un fondo che noi volevamo

che vuole rendere tutto sempre più difficile; vogliamo garantire il diritto anche delle persone del Nord di potersi muovere? Perché mi sembra che le tasse le paghiamo, e abbondantemente. Vi è Vi è un'evidenza in questo Paese: le spese per la pubblica amministrazione stanno galoppando sempre più forte e tutti i provvedimenti che avete messo in finanziaria per cercare di contenerle sono lettera morta. In un periodo in cui si parla degli stipendi della politica, la finanziaria pensava di tagliare un dieci per cento degli stipendi dei *manager* dei Ministeri, che non sono pochi.

accertati di fronte alla giustizia tributaria rispetto ai primi sei mesi. Prima decidete con gli studi di settore quanto i liberi professionisti devono versare, e lo decidete immancabilmente, minacciando eventuali controlli; dopo - solo dopo - date al contribuente l'onere della prova contraria. Questo contrasta con il diritto dei contribuenti e contrasta anche con il buonsenso: andate a tosare sempre gli stessi e vi dimostrate, quindi, forti con i deboli e molto deboli, invece, con i forti. Alle moschee, che ormai - mi sembra evidente - sono soggette ad una forte infiltrazione terroristica, vengono dati soldi. Abbiamo proposto di controllare le false pensioni INPS. Ci sono italiani che continuano a riscuotere la pensione dei genitori (qualcuno è assurto agli onori della cronaca perché era nel congelatore), ma abbiamo trovato fatti concreti di evasioni di extracomunitari, che hanno genitori al paesello di 115 o 116 anni e che continuano a riscuotere la pensione. Questo è un tesoretto che non volevamo condividere nel Parlamento. Il tesoretto è dei contribuenti e dei cittadini padani, del centro e meridionali, è il frutto delle tasse che avete tagliato e che avete imposto ai contribuenti. Per questo voteremo contro, per questo siamo fortemente contrari:

Signor Presidente, le ragioni del voto favorevole di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea in merito sono state esposte dal collega Tecce, quindi mi soffermo soltanto su alcune considerazioni.

di essere conservatori e reazionari perché difendiamo i lavoratori dipendenti, i pensionati, i giovani precari e così facendo non ci renderemmo interpreti dei processi di modernizzazione, delle magnifiche sorti progressive che possono venire al Paese dal picchiare sodo sui pensionati e sui giovani precari, accontentando così Almunia e vari altri eurocrati, a cui sembra doversi confermare quotidianamente una sorta di reverenza. noi siamo stati impegnati a trovare delle soluzioni minimali e a partecipare anche alla costruzione di soluzioni impegnative

ma come non valorizzare il fatto che, a proposito della tassazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti (i cosiddetti studi di settore), a fronte anche, come dire, di qualche superficialità, qualche improvvisazione o magari disattenzione da parte del Governo e dell'amministrazione (che avrebbe dovuto dare seguito al protocollo del dicembre 2006 con le associazioni),

e poi una soluzione concordata e contrattata con il Governo, filtrata attraverso la ripresa del confronto tra il Governo e le associazioni imprenditoriali, e che ha dato luogo

tant'è che le previsioni della legge finanziaria assegnate agli studi di settore vengono confermate, malgrado la normativa non fosse particolarmente adeguata. luogo, perchè, attraverso quel confronto, siamo arrivati a dare degli studi di settore e degli indici di normalità un'interpretazione che, per un verso, mette i contribuenti nella condizione di essere garantiti rispetto all'amministrazione e, per altro verso, mette l'amministrazione nella condizione di

dall'altra, con la revisione della normativa sugli studi di settore, in particolare sugli indici di normalità, così noi possiamo prepararci, alla luce del DPEF approvato

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario (che ha avuto la pazienza di seguire questo dibattito sin dall'inizio) vogliate nei limiti in cui vi è dato e desiderate farlo - delle motivazioni che indurranno Forza Italia a votare negativamente su questo provvedimento comunemente detto «dell'utilizzo del tesoretto». Le motivazioni possono essere così sintetizzate. Il provvedimento non evidenzia una virulenza, un piglio ed un impegno di pari intensità e rigore, a livello di spesa pubblica, di quello più volte enunciato con riferimento al recupero della cosiddetta evasione fiscale. Ed è appena il caso di dire che non ci potete trovare d'accordo quando dite che le maggiori risorse provengono dalla paura che il Governo, con il suo eccessivo conclamato e dichiarato rigore, ha voluto incutere al contribuente, ai ceti produttivi che evidentemente si sarebbero determinati a pagare più imposte e tasse. Non è stato proprio così.

che i provvedimenti proposti e adottati da questo Governo nel corso di appena un anno di gestione abbiano potuto determinare il cosiddetto tesoretto. Il cosiddetto tesoretto viene dalla virtuosità delle politiche praticate nel corso dei cinque anni del Governo Berlusconi, che ha anteposto l'interesse del sistema produttivo all'interesse dello Stato, della pubblica amministrazione, molto spesso incline a prediligere la spesa corrente rispetto alla spesa per investimento. Tornando alle motivazioni sinteticamente esposte, non vi è stato un *animus* corrispondente a quello che avete dichiarato di voler esercitare a livello di entrata con riferimento alla spesa. Ed è sufficiente poi totalizzare le spese che deriveranno da questo provvedimento, tra spesa corrente e spesa per investimento, per rendersi conto che chi la fa da padrone è la spesa corrente.

perché continuando ad usare i tesoretti, per buona parte ai fini della spesa corrente, questo Paese non solo non persegue, ma nemmeno conseguirà risanamento. Per questi motivi, evidentemente, dichiariamo il nostro voto contrario al provvedimento.

prima di sviluppare alcune riflessioni, vorrei chiosare alcuni interventi che ho ascoltato, in particolare per segnalare un approccio che mi pare significativo della discussione rispetto al provvedimento in esame. Ritenevo che ci trovassimo di fronte ad un contesto europeo

si delineava un maggiore *stock* di entrate e che quindi vi fossero dei fenomeni importanti, significativi su cui porre l'attenzione, sia rispetto alla precedente attività del Governo di centro-destra sia rispetto allo scenario all'interno del quale noi viviamo, per cercare di individuare alcuni elementi significativi, non solo relativi al sistema Paese. Invece, dal dibattito e soprattutto da alcuni interventi, mi sono reso conto che le cose sono molto più tranquille e semplici, cioè a dire, se di fronte a maggiori entrate ci troviamo, tutto questo non dipende da un'attività di Governo,

che il centro-sinistra continua ad avere nel tentativo d'interpretare la realtà non per quello che essa esprime, manifesta, evidenzia, ma sulla base di un assunto ideologico. Fatta questa

qual è l'idea dell'Italia che si ha e qual è l'idea della modernizzazione italiana che si vuole concretizzare e realizzare. La sinistra un'idea non ce l'ha, non declina il futuro e ripete alcune forme del passato, fuori tempo e fuori dal tempo; è politicamente e socialmente autoreferenziale, arroccata nella torre eburnea della maggioranza e minoranza e della rappresentazione sociale e delle forme della rappresentanza sociale della vecchia Italia; riscrive pensioni e *welfare*, non per ridefinire il patto generazionale, ma per tenere e mantenere il patto politico di maggioranza e di alleanza sociale sociale con la vecchia Triplice, senza autonomi, senza professionisti, senza giovani, per tutelare il vecchio cartello dei garantiti. In fondo, questo provvedimento è tutto dentro questa impostazione culturale.

che già di per sé è un elemento che ha determinato per la prima volta l'utilizzo del salario differito per finanziare opere pubbliche, introducendo un meccanismo all'interno della finanziaria quantomeno discutibile, ed oggi si arriva all'anticipazione di cassa nell'attesa che si determinino le entrate, quindi a un provvedimento che trova copertura senza che ancora si realizzi l'assestamento di bilancio, per cui si determina un meccanismo che vede prima le spese e poi la certezza delle entrate. Ho citato il trattamento

che determina uno squilibrio ulteriore, anzi un paradosso, per cui sostanzialmente la svalutazione competitiva la fanno i settori forti dell'industria dell'industria e sul piano territoriale determinando un'ulteriore sperequazione per il Mezzogiorno, nel Documento di programmazione economico-finanziaria non avete voluto nemmeno approvare un'indicazione relativa alla negoziazione, in sede europea, della fiscalità compensativa per il Mezzogiorno, che invece è un elemento che dovrebbe accompagnare la riflessione sull'impatto

provvedimento, nel determinare le condizioni di accesso a questo presunto fondo dirigista gestito dal Ministero rappresentato

il provvedimento oggi in discussione riguarda la conversione del decreto-legge in merito all'uso e alla ripartizione di quella quota di extragettito fiscale ai più nota col nome di «tesoretto». Un argomento che ha rappresentato il «tormentone» pre-estivo di questi ultimi mesi e che Prodi e compagni hanno provato ad utilizzare come specchietto per le allodole per fare credere agli italiani che il «gruzzolo» che lo Stato si è ritrovato inaspettatamente in tasca fosse il frutto delle incredibili politiche economiche di questo Governo. La verità, colleghi, la conosciamo tutti. Alla fine del 2006 questo Governo ci faceva dono della finanziaria. Un provvedimento che ha paralizzato interi comparti produttivi e ha prelevato fior di miliardi dalle tasche degli italiani sotto il nobile obiettivo di ridurre il debito pubblico, ma di fatto mettendo spalle al muro il nostro Paese. Cosa ancor più grave è che mentre le famiglie italiane si barcamenavano per riuscire a raggiungere fine mese e le nostre imprese arrancavano sotto l'imposizione di nuove tasse, il vostro zelante Governo si accorgeva di un particolare di non poco conto: forse i soldi prelevati erano troppi. E a questo punto, invece di utilizzare il disavanzo di cassa per il risanamento dei conti pubblici, cosi come auspicato da tutte le principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali, eccoci qui a discutere delle elargizioni a pioggia fatte con questo decreto-legge. Prodi, infischiandosene dei moniti del Governatore della Banca d'Italia, della Commissione europea, del Fondo Monetario Internazionale, ha deciso di utilizzare il disavanzo di cassa per ridare una boccata di ossigeno al Governo che aveva ormai consumato tutta la sua riserva. Quindi, via le buone intenzioni, altro che debito pubblico e largo ad una serie di microinterventi settoriali che non servono al bene del Paese, ma a saziare i perenni appetiti della sinistra comunista. Il Governo Prodi, dopo mesi di ricatti, colpi di mano e richieste più o meno velate, ha utilizzato questo inaspettato *surplus* elargendo «contentini» di chiara matrice ideologica, ma lasciando irrisolti i veri problemi del Paese. Un Governo coscienzioso che si fosse trovato fra le mani un extragettito non avrebbe nemmeno preso in considerazione la possibilità di trattarlo come un patrimonio al di fuori della contabilità ordinaria, ma lo avrebbe immediatamente impiegato a copertura del *deficit* statale. Colleghi, l'extragettito meritava una destinazione diversa, una destinazione volta al riequilibrio del sistema economico e alla riconsegna indiretta ai cittadini di quanto gli è stato indebitamente tolto attraverso l'utilizzo della leva fiscale. così come fatto con la finanziaria e con il DPEF appena approvato, vi siete più preoccupati di accontentare coloro che politicamente vi sono vicini, dimenticandovi distrattamente o volutamente dei grandi problemi economici, industriali e sociali del nostro Paese. Mossi da logiche clientelari, ci proponete oggi una serie di misure di breve respiro, dimostrando ancora una volta l'assenza di un disegno strategico, trascurando le esigenze generali ed in particolare del Sud e delle nostre isole, dalla Sicilia alla mia Sardegna, marginalizzate nel contesto italiano e tenute staccate da tutte le dinamiche economiche e sociali del resto del Paese più evoluto. Colleghi, questo decreto-legge che per rilevanza ed entità delle misure previste rappresenta una sorta di minifinaziaria aveva l'obbligo di fare di più! Aveva l'obbligo di interessarsi delle mancanze del sistema sicurezza, dell'università, della ricerca e addirittura del comparto primario, l'agricoltura, che viene invece totalmente snobbata e messa in forte difficoltà con politiche deboli ed inefficaci. Al presidente Prodi dico che non occorre prodigarsi molto per evidenziare tutte le contraddizioni di questo Governo. Un Governo che promette ma che di fatto non fa nulla di concreto. A cominciare dalle 281 pagine del programma elettorale, dal pomposo ed ironico titolo «Per il bene dell'Italia», in realtà alla fine solo carta straccia. E che dire dei 12 punti per il rilancio dell'azione di Governo, un documento che si poneva un unico obiettivo: quello di far restare in sella questo Governo e questa maggioranza dopo lo scivolone sulla politica estera. A questo vanno aggiunti la fasulla riforma dell'ordinamento giudiziario, il pasticciato accordo sulle pensioni e l'illusorio Documento di programmazione economica-finanziaria approvato la settimana scorsa. Per un anno avete sostenuto che il Governo Berlusconi aveva lasciato una voragine nelle casse dello Stato e poi siete stati stati puntualmente smentiti non appena sono giunti i primi rendiconti annuali. Per un anno avete sbandierato il risanamento dei conti pubblici, obiettivo cardine della vostra ultima legge finanziaria, salvo poi accantonarlo accantonarlo alla prima occasione concreta. Tutto si scioglie come ghiaccio al sole, quindi. L'unica certezza è che in poco più di un anno di governo siete riusciti a dilapidare le risorse del Paese, a bloccare la crescita economica, a far riprendere l'indebitamento e nonostante tutto, consentitemi

imponendo la ventesima fiducia in un anno, il Governo istituisce qui a Palazzo Madama la scelta, quasi sicura, del prendere o lasciare proponendo un documento immodificabile e umiliando di fatto il ruolo del Senato quale rappresentante delle istanze del popolo italiano. la politica di questo Governo è devastante per il Paese, ma fortunatamente gli italiani se ne sono già accorti.

ragioni e delle riflessioni che il Gruppo dell'Ulivo fa in questo dibattito e su questo provvedimento. Il mio intervento sarà diviso in due parti: nella prima, brevissima, mi riporterò

dire poco fa, ma importanti e strategiche per l'interesse e lo sviluppo dell'economia italiana e per rispondere alle domande che dalla società italiana sono emerse anche nel dibattito *post* finanziaria, cioè nella discussione che c'è stata dopo l'approvazione della legge finanziaria. Cito soltanto gli aspetti più importanti: la norma in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali, che non è tutto quello che gli enti locali desideravano, ma certo dà una risposta ad uno dei problemi più gravi; l'aumento delle pensioni basse, anche questo uno degli obiettivi che noi ci eravamo dati e che con questo provvedimento, sia pure non nella misura in cui sarebbe necessario, incominciamo ad attuare; l'attribuzione di risorse ad ANAS e Ferrovie per gli investimenti; la modifica della normativa in materia di studi di settore, accogliendo le richieste delle categorie del

di programmazione economico-finanziaria e già allora noi avevamo spiegato che, con il provvedimento contenuto nel decreto-legge n. 81, avremmo fatto un intervento di sviluppo ed equità, dopo una finanziaria dura, e avremmo posto posto le basi di una manovra espansiva finalizzata a consolidare la crescita. Queste le ragioni di merito. Tuttavia (e inizia qui la seconda parte del mio intervento leggermente più ampia della prima), non voglio sottrarmi alla discussione, prevalente in quest'Aula,

avanzata da molti colleghi, sostiene che il provvedimento è finanziato in *deficit* e che peggiora i saldi di finanza pubblica. Vorrei invitare i colleghi a rivedere l'articolo 1 del decreto, che ora leggo sinteticamente: «Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali (...) sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica (...) definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008- 2011». Ricordo che il Documento di programmazione economico-finanziaria prevedeva

Quindi, non vi è nessun finanziamento in *deficit* e nessun peggioramento dei saldi di finanza pubblica, ma un rispetto dei saldi del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La nostra posizione, illustrata dal relatore Ripamonti, prevedeva che le maggiori entrate strutturali potessero essere utilizzate per finanziare maggiori spese, mentre le maggiori entrate derivanti dal ciclo economico non strutturali dovessero essere destinate all'abbattimento del debito e al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

documento del Servizio del bilancio del Senato, ricostruendo questo calcolo, arriva alla conclusione che fondamentalmente lo 0,3

siamo molto tranquilli sul piano dei problemi affrontati e sappiamo di aver indicato soluzioni significative per problemi importanti del nostro Paese.

e, come ho avuto modo di dire in quel ramo del Parlamento, il Governo con questo decreto, cui attribuisce una grande importanza, ha inteso proseguire nella direzione indicata fin dall'inizio della legislatura, da una parte, un'azione di risanamento forte e necessaria e, dall'altra, l'attuazione di misure altrettanto necessarie per l'equità sociale e il sostegno allo sviluppo.

aveva certificato uno sfondamento nell'equilibrio tra *deficit* e prodotto interno lordo che rendeva necessaria una manovra di risanamento che avrebbe dovuto portare quest'anno - come è avvenuto

il rapporto tra prodotto interno lordo e *deficit* al 4,1 per cento era stato reso possibile da un decreto che il Governo di centro‑sinistra aveva dovuto emanare (uno dei primi atti di Governo) nel luglio dello scorso anno, in cui era stato disposto un intervento rilevante sui conti

per raggiungere quest'obiettivo, siamo stati contestati dall'opposizione rispetto a questo punto, cioè alla necessità di misure rigorose e forti per rientrare all'interno del patto di stabilità con l'Unione Europea. Sento stasera e ho visto in questi giorni - vi è stato anche alla Camera dei deputati - che, viceversa, l'opposizione rimprovera il Governo e la sua maggioranza

realizzato, ma migliorato perché il *deficit* annuale è del 2,1 per cento. Vi è stata una discussione con l'Unione Europea e noi riteniamo

allo stesso tempo, di utilizzare una parte di risorse, lo 0,4, per poter dare forza anche a quegli aspetti di equità e di sostegno allo sviluppo, senza cui un Paese non cammina e non raggiunge neppure in modo consolidato alla lunga Questa è la scelta che sta dietro alle misure che noi abbiamo assunto. Tra le misure contenute in questo decreto, voglio ricordare in particolare - è stato fatto ora

e l'anticipo che verrà dato a settembre a oltre tre milioni di cittadini, senza che questo incremento di reddito sia sottoposto a tassazione.

muoversi in questo Paese per vedere qual è la condizione di vita di alcune famiglie, soprattutto di quelle che hanno redditi di pensione molto bassi. Tuttavia, è una misura concreta che va in direzione dei ceti che hanno la possibilità da parte di Province e Comuni di utilizzare gli avanzi di amministrazione, siamo solo parzialmente soddisfatti, perché nel Patto di stabilità costruito - a dir la verità è stato concordato anche con le associazioni dei Comuni e delle Province

La misura presa va nella direzione giusta, anche se è parziale e questo è un punto che dovremo nella legge finanziaria sottoporre ad un confronto, ad una valutazione e ad un approfondimento serio per vedere di migliorarlo e correggerlo.

riscatto della laurea in modo più agevolato; le risorse messe a disposizione per la sicurezza e per gli stessi Vigili del fuoco;

del riferimento anche agli indicatori di normalità economica. Voglio, tra l'altro, sottolineare, da questo punto di vista, che su questo tema

un sostanzioso contributo al Fondo per la lotta contro l'AIDS, l'incremento dei trasferimenti a poste, ferrovie, ANAS ed ENAV. E per lo sviluppo - ultima considerazione che voglio fare - vi è la riduzione delle tasse sul lavoro e il fatto che questa avvenga in modo più accentuato, doppio, per il Mezzogiorno, così come lo sblocco degli interventi per il Mezzogiorno, ad esempio sulla legge n. 488, e la possibilità di intese anche di settore. Comunque, per quanto riguarda il Mezzogiorno, voglio dire che il Governo ha assicurato una serie di risorse di compartecipazione nazionali e regionali, nonché politiche comunitarie che fanno sì che il Mezzogiorno abbia il problema, se vogliamo essere seri, di selezionare bene gli obiettivi e i programmi che vuol portare avanti. Non c'è una questione di mancanza di risorse realizzare, c'è la necessità che questi programmi e obiettivi siano effettivamente tali da poter essere realizzati, da poter dare un contributo ai cittadini allo sviluppo di queste aree e fare in modo che, magari nel 2013 (dato che queste risorse sono a disposizione da qui al 2013), in Europa, come oggi si dice: «Guardate come sanno spendere bene i fondi l'Irlanda o la Spagna», si possa dire: «Guardate questi fondi che erano stati programmati come sono stati spesi con efficacia e per obiettivi giusti nel Mezzogiorno d'Italia». So bene che il tempo a disposizione del Senato è stato contenuto, anche se ciò, come ho cercato di ricordare, non significa che il Parlamento nel suo insieme non abbia avuto tempo per esaminare il provvedimento e che non ci sia stato un confronto nel corso di questi mesi. Una parte di quanto facciamo era negli impegni che abbiamo assunto quando abbiamo discusso della legge finanziaria. Sono anche consapevole del fatto che in un sistema bicamerale paritario, a volte, la Camera che affronta il provvedimento in seconda lettura ha vincoli di tempo più stringenti. Per l'ordinamento giudiziario, per fare un esempio concreto e recente, è stata la Camera dei deputati a doversi muovere in orizzonti temporali e di contenuto maggiormente condizionati. Questo decreto, comunque, nel testo approvato alla Camera, lo ripeto, tiene conto di un confronto che si è svolto nel corso degli ultimi mesi, prima, con e dopo la finanziaria. Tiene conto del fatto che per il Governo è un punto fermo proseguire sulla strada sulla strada che tenga insieme consolidamento del risanamento dei conti, e, al tempo stesso, capacità di rafforzare in modo coerente politiche di equità e sviluppo.

io assumo, con chiarezza, a nome del Governo, la responsabilità di varare questo provvedimento senza modificarne gli equilibri, per il valore che per noi hanno e per la necessità di farli entrare in vigore subito.

Vorrei ricordare che al Senato, negli ultimi quattro mesi, ci sono stati almeno due dibattiti di politica estera ed è stato esaminato il DPEF. Quindi, non importa fare questo tipo di polemiche, che non hanno fondamento. In questo caso, non ci sono ostruzionismi, né altro: il Governo si assume la responsabilità di chiedere la fiducia - ripeto perchè, per il valore che questi contenuti hanno, non sarebbe giusto modificare gli equilibri delle scelte poiché vi è la necessità di farli entrare in vigore subito, altrimenti lo stesso anticipo delle pensioni minime a settembre non vi potrebbe essere. Per queste considerazioni, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi,

dell'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento da parte del Governo. Conformemente alla prassi, trasmetto il testo del provvedimento alla 5a Commissione permanente, perché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria

sulla questione di fiducia, che dovrà concludersi entro le ore 14 al massimo, con tre ore assegnate all'opposizione e un'ora e mezza alla maggioranza. Ove la discussione generale si concludesse prima delle ore 14, potremo avviare le dichiarazioni di voto in modo da arrivare, intorno alle ore 14,30, al voto di fiducia.